L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

ne è seguito ha dimostrato chiaramente quanto io stesso avevo detto nella parte conclusiva della mia relazione. Negli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione - che tutti ringrazio - si è compreso con grande chiarezza che, pur nella diversità di vedute su alcuni aspetti, pur con le critiche che vengono mosse su alcune sue parti, in realtà

è stato fatto, senza pregiudiziali politiche, nel tentativo di dare un buon provvedimento al nostro Paese. Comprendo che ragioni politiche di natura generale, che possono forse riguardare questioni più ampie che non questo provvedimento, possono portare ad atteggiamenti d'Aula nel voto finale che nella loro rappresentazione formale finiscono per tradire sostanzialmente la

non avendo mai ritenuto di mettere piede per un solo minuto nell'Aula delle Commissioni che si sono occupate per mesi di questo provvedimento,

e ringraziando anche per il ritiro di alcuni emendamenti che vengono trasformati in ordini del giorno, concludo la replica ringraziando ancora tutti quelli che hanno contributo alla redazione del testo che questa mattina diventerà legge della nostra Repubblica.

Ricordo che questo provvedimento è stato approvato in Consiglio dei ministri come collegato alla finanziaria triennale nel giugno dello scorso anno. È subito approdato a questa Camera a questa Camera e qui penso si sia svolto, senza nulla togliere all'altro ramo del Parlamento, il lavoro più intenso e importante. Ricordo il lavoro del Comitato ristretto

Il lavoro è stato condotto in maniera trasparente, onesta e con la volontà da parte del Governo di migliorare il testo sentendo le opposizioni e soprattutto quanto di meglio la cultura giuslavoristica e aziendalistica italiana e non solo aveva prodotto nel settore in

C'è stato un approfondimento, che fra l'altro verrà recepito da un ordine del giorno, attraverso il quale in maniera innovativa il Governo accetta di

ancora. È relativamente facile scrivere un testo di legge, è relativamente facile scrivere decreti legislativi: la cosa più difficile è poi realizzare quanto ci si è impegnati a fare con una legge, e quasi sempre le nostre leggi sono carenti da questo punto di vista. Il Governo si impegna

perché inizia un processo, una piccola grande rivoluzione, un piccolo grande cambiamento che modificherà la vita di 60 milioni di cittadini italiani nel senso dell'efficienza, della trasparenza, della responsabilizzazione. Ricordiamo che questa riforma

Senza una pubblica amministrazione efficiente, non si fa una scuola efficiente, non si fa una giustizia efficiente, non si fa una sicurezza efficiente, non si fa una politica economica efficiente. In altre parole, lo Stato non è efficiente. Il cittadino deve essere al centro delle attenzioni della pubblica amministrazione, cosa che non è mai avvenuta in questo Paese. Stiamo iniziando un percorso nuovo che ha bisogno di tutti e ha bisogno certamente dell'attenzione, del controllo e del consenso del Parlamento. Fin dall'inizio ho esplicitato questa volontà e penso di essere stato Mi dolgo che non vi sia un voto favorevole da parte dell'opposizione. Posso capire le ragioni politiche. Credo però che il lavoro comune che dovremo fare con i decreti delegati e nella verifica dello stato di implementazione possa vedere l'opposizione partecipe. Ancora grazie Ancora grazie al Senato della Repubblica, grazie al relatore e a tutti coloro che hanno lavorato, grazie all'opposizione, grazie all'intero Parlamento.

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, lettera *g)*, avvenga nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio destinate all'attività di formazione e che l'integrazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 4, costituisca una mera facoltà

a concorrenza di fonti, tra fonte legislativa e fonte contrattuale, si determini una sovrapposizione del contratto collettivo rispetto

immediatamente e direttamente desumibile dai princìpi generali dell'ordinamento; riteniamo non sia necessario precisarlo. In

di una incapacità del *management* pubblico di gestire l'autonomia collettiva con il dovuto rigore e con la dovuta coerenza rispetto alle linee di buona gestione dell'amministrazione.

stimolare e a garantire l'impegno del *management* pubblico, cui è affidata la contrattazione collettiva, affinché la sua funzione sia gestita in modo più rigoroso e più efficiente rispetto al passato. In quel modo non ci sarà più bisogno di interventi legislativi correttivi e si ripristinerà - e avrà pieno corso - quel principio del contrattualismo che tutti riconosciamo, e abbiamo sancito anche in questo testo legislativo, come il principio ispiratore dell'intero sistema.

il ragionamento fatto dal collega Ichino e riteniamo che l'articolo in esame sia complessivamente peggiorativo dell'intero impianto della norma. all'interno di esso si aggiungono discrezionalità e comunque interpretazioni tali da rendere assolutamente confusa un'applicazione allorquando - come diceva il collega Ichino - si succedano nel tempo diverse fonti

In tutti i Paesi che hanno adottato il principio della trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche in particolare mi riferisco al *Freedom of Information Act* statunitense ed al *Freedom of Information Act* britannico, entrambi ispirati alla legge svedese della metà degli anni '70 informazioni attinenti al rapporto di lavoro, con esclusione soltanto delle notizie sensibili (quindi quelle

delle retribuzioni, tutte le vicende del rapporto di lavoro, comprese le sanzioni disciplinari, all'assenza per malattia, il dato che viene reso accessibile è il dato aggregato per ufficio. Per quanto riguarda le valutazioni del preposto, del responsabile dell'ufficio, l'orientamento è di rendere accessibili quelle valutazioni individuali riferite a singoli professionisti - come ad esempio i singoli magistrati nell'esercizio della loro funzione, i chirurghi, gli alti funzionari - nel caso in cui l'attività del singolo è attività della funzione, mentre a livello inferiore l'orientamento prevalente e migliore è quello della valutazione aggregata del *team*, della singola squadra. la scelta sul tipo di valutazione, e quindi di informazione, sarà compiuta dall'agenzia centrale, che dovrà impartire direttive di carattere generale, a cui si atterranno naturalmente gli organi di valutazione inferiore. Tutto questo è precisato nell'ordine del giorno accolto dal Governo e credo che sarà bene venga precisato con altrettanta chiarezza nei decreti delegati che seguiranno.

un arricchimento molto opportuno della normativa in esame, perché tende ad enfatizzare e valorizzare i processi di mobilità sia volontaria che non, anche

in una situazione qual è quella delle amministrazioni pubbliche in generale e in particolare dell'amministrazione statale, dove i processi di mobilità

Ora, siamo pienamente d'accordo che, quando si tratta di trasferire una persona da una città all'altra, il trasferimento debba essere volontario, altrimenti si trasforma in un licenziamento,

trasferimento all'interno dell'Amministrazione del lavoro tra addetti ai servizi di collocamento alla direzione del lavoro e ispettorati. vi è sovrabbondanza di personale addetto agli uffici preposti ai servizi per l'impiego, vi è grave carenza agli ispettorati se assegnassimo uno o due segretari o assistenti per ogni ispettore si potrebbe moltiplicare per due o per tre l'attività degli ispettori.

qualsiasi buona organizzazione deve poter operare trasferimenti di questo tipo, anche unilateralmente. Se non entriamo in questo ordine di idee, continueremo ad avere zone di gravissimo spreco e zone di sofferenza nell'efficienza dell'amministrazione pubblica. È questo uno dei punti in cui maggiormente si nota l'effetto negativo dell'abdicazione del *management* pubblico alle proprie funzioni. Quindi, ritengo sia particolarmente importante che venga recuperato recuperato questo potere. Quando ieri ho parlato della tenaglia del circolo vizioso della irresponsabilità, mi riferivo anche e soprattutto a questa materia.

Signor Presidente, la questione dell'organo indipendente di valutazione ha una sua Abbiamo seguito il tentativo di definirla in maniera soddisfacente, ma alla fine non possiamo dirci soddisfatti. Siamo convinti che sarebbe stato meglio istituire una commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche sulla base di quella già prevista nella scorsa legislatura all'interno del disegno di legge di iniziativa dell'ex ministro Nicolais e approvata, peraltro, dalla Camera dei deputati. Il problema è che, così come si configura la commissione di valutazione nel testo attuale, si ha un organismo all'interno dell'ARAN che, di fatto, non garantisce una posizione indipendente.

Inoltre, dobbiamo osservare che questo organismo, composto da cinque membri che non hanno un'esclusività di rapporto, è dotato di un fondo spropositato rispetto ai compiti. È vero che l'indipendenza costa,

il Gruppo dell'Italia dei Valori esprime contrarietà alla definizione specifica di questo organismo centrale, non all'idea Non ci convince il modo in cui è stato pensato. Non ci convince l'enormità della spesa destinata a questa funzione.

giugno 2008 quando il signor ministro Brunetta affermò testualmente a Radio R101: «Stiamo studiando una grande innovazione, che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio: applicare la *class action*, che stiamo riscrivendo, anche per il settore pubblico. I cittadini potranno arrabbiarsi, utilizzando le associazioni dei consumatori, fare causa a quei settori della pubblica amministrazione che non funzionano e vederli condannati».

affermava: «Si sta discutendo di come migliorare l'efficacia e la trasparenza della norma» anche per poterla estendere alla pubblica amministrazione. Signor Ministro, lei chiede fiducia. Ma quale fiducia può avere nel Governo quel milione di risparmiatori frodati

inserire nella normativa l'istituzione di un reato, prevedere l'irrogazione di una pena, però nella pubblica amministrazione non può valere.

non in riferimento alla media, come normalmente accade nei Paesi in cui questo metodo viene applicato, ma addirittura alla media del quartile più alto, vale a dire sostanzialmente a quella della testa della graduatoria. Un obiettivo di questo genere, che significa che la centesima amministrazione sarebbe obbligata ad allinearsi alle prime, è evidentemente impossibile, quindi inesigibile. Si tratta della classica norma "fuga in avanti", che serve a ridicolizzare il metodo del *benchmarking* perché, laddove la cosa è palesemente inesigibile, quella cosa non si farà

l'emendamento 4.11 è stato trasformato), che riconduce il discorso nei termini di una logica gestione del metodo del *benchmarking*, che implica anche una sua flessibilità e una sua ragionevolezza. Saranno poi gli organi politici, nel fissare gli obiettivi alla dirigenza apicale, e la dirigenza apicale, nel fissarli alla dirigenza inferiore, ad individuare l'obiettivo esigibile, in quanto effettivamente realizzabile, che possa veramente agire da stimolo ed incentivo.

ripeto ancor una volta, fino alla noia, che non è possibile che il Governo affermi di voler tutelare i cittadini

una cosa che non dovrebbe essere più ricordata, cioè che ciascuno dovrebbe votare per sé. Prego i senatori Segretari di provvedere al ritiro di tutte le tessere

Signor Presidente, l'emendamento è inteso a dimezzare i costi dell'organismo centrale, di cui al comma 2, lettera

con l'approvazione di un emendamento del Governo, con il quale si intende sprecare 4 milioni di euro per il finanziamento di non meglio specificati progetti sperimentali ed innovativi, decisi con decreto interministeriale dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Il 4.8 è quindi un emendamento rivolto ad una attività virtuosa di risparmio.

Con questo emendamento si propone che vengano rispettate le norme a tutela delle persone, in particolare della *privacy*, chiamando in campo il garante per la protezione dei dati personali. Non vorremmo che venissero violate le leggi che esistano in questa materia e crediamo che sia opportuno inserire questa minima garanzia, pur dando atto della necessità di una trasparenza su questa tematica. Chiediamo quindi che l'accesso alle notizie che riguardano lo svolgimento di prestazioni di soggetti addetti a funzione pubblica

raccomanda, anzi vincola il Governo ad attribuire un peso decisivo, tra i criteri per la nomina dei membri della commissione centrale, a quello commissione centrale, a quello dell'acquisizione di un'esperienza pluriennale acquisita in organi indipendenti di valutazione della produttività ed efficienza di amministrazioni pubbliche e private in particolare in Paesi stranieri. A mio avviso, questo punto è particolarmente rilevante perché sul terreno della cultura e della pratica - della buona pratica - della valutazione nelle amministrazioni pubbliche il nostro Paese, se non è all'anno zero, è all'anno 0,1: siamo molto, molto indietro rispetto a Paesi che praticano la valutazione e ne hanno affinato i metodi attraverso decenni di esperienza.

Per questo credo sia importantissimo che noi utilizziamo, nell'agenzia creata a livello centrale, persone che portino in Italia la migliore esperienza dei Paesi nordeuropei. chiedo che su questo punto ci sia un voto di conferma del Senato.

non solo il modestissimo sottoscritto, ma altri colleghi hanno tentato di concretizzare in prima lettura e che - di ciò me ne compiaccio - con uno sforzo congiunto della maggioranza, del Governo e dell'opposizione si concretizza in questo momento. Si tratta di una norma equilibrata e di una mediazione accettabile; resta il rammarico che questa facoltà, che è prevista a beneficio dei dirigenti della struttura complessa del Servizio sanitario, non si sia potuta estendere anche ai dirigenti delle strutture semplici o ai titolari di incarichi professionali. Ciò sarebbe stato oggettivamente più equo, tenuto presente soprattutto che in tutte le Regioni molte ASL stanno applicando questa norma in maniera discutibile e, in qualche caso, forse settaria. Ciò è molto odioso nei confronti di professionisti che operano nelle nostre strutture ospedaliere e sanitarie. Ritengo che abbiamo fatto una cosa molto importante trovando una mediazione avanzata

sarebbero stati nella condizione di dover necessariamente lasciare il loro lavoro, con una disparità di trattamento, ai limiti della incostituzionalità, tra chi aveva versato una contribuzione figurativa e chi aveva invece maturato un'effettività

Signor Presidente, come taluni colleghi avranno la bontà di ricordare, in prima lettura, insieme al senatore Izzo e ad altri colleghi del Gruppo, abbiamo cercato di dare un contributo alla soluzione positiva

Il punto, onorevoli senatori, è il seguente. Possiamo dare una risposta affermativa o negativa alla questione della vicedirigenza e al problema dei quadri nel pubblico impiego, questione che nel privato è ampiamente risolta in un certo senso.

se debba esistere un istituto di vicedirigenza o di quadri con determinate responsabilità e funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione, poiché questa è una decisione propria della pubblica amministrazione e dello Stato nei suoi ambiti esecutivo e legislativo.

Che lo si debba rimettere totalmente ad una decisione o codecisione di carattere sindacale mi sembra inopportuno. Fermo restando che le applicazioni e le articolazioni debbono certamente essere negoziate con le organizzazioni sindacali, che sicuramente offrono un contributo di esperienza

Presidente, comprendo le ragioni che hanno ispirato gli emendamenti del senatore Benedetti Valentini, che peraltro sono stati oggetto di dibattito sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Naturalmente, signor Presidente, come lei mi insegna, nel glossarietto parlamentare gli ordini giorno, in ordine alla loro efficacia decrescente si distinguono in grida manzoniane, farfalle sotto l'Arco di Tito, meri auspici e pie intenzioni. non vorrei iscrivermi ad alcuna delle quattro categorie, ma più modestamente avere dal Governo il proponimento di riesaminare e riprendere in considerazione le valutazioni di opportunità in ordine a questa tematica, sia nel dialogo con le organizzazioni sindacali sia nelle proprie determinazioni, perché sia riportata ad una normativa organica la decisione dei caratteri fondamentali dell'istituto, fermo restando che le articolazioni pratiche sono largamente rimesse alla interlocuzione della contrattualistica collettiva nazionale.

fornisce una lettura meramente interpretativa dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di vicedirigenza, impegna il Governo a riprendere in esame, nei tempi più ravvicinati possibile, l'intera problematica della istituita vicedirigenza, facendosi promotore di una sistemazione normativa organica che stabilisca i caratteri fondamentali dell'istituto nell'interesse proprio e generale della Pubblica Amministrazione,

Signor Presidente, è per me fonte di grande imbarazzo intervenire - lo faccio per dovere istituzionale - essendo a tutti nota l'amicizia profonda e la stima autentica che mi lega al collega Benedetti Valentini.

improprietà organizzativa, che tra l'altro è ancora più nitidamente tale se comparata alla vanità nella quale è scivolata la norma, che aveva a sua volta, per il settore privato, istituito la categoria dei quadri. Si tratta di ridondanze organizzative che diventano soltanto sacche per elementi di gestione non limpida, non trasparente, non efficace, non capace di modularsi flessibilmente sulle esigenze che competitivamente emergono. Non a caso il testo che oggi viene sottoposto all'Assemblea è frutto di una mediazione attenta, intelligente e prolungata che sostanzialmente, lasciando alla libera determinazione delle parti sociali l'introduzione della vicedirigenza, può tenere conto dei casi nei quali si manifestino condizioni così specifiche e articolazioni così disallineate rispetto alla media del settore pubblico da meritare una risposta organizzativamente rilevante su questo versante. Mi sembra già una concessione ampia e significativa, ragion per cui andare oltre, cioè impegnare il Governo

Con l'articolo 9 si vanno ad attribuire ulteriori funzioni al CNEL, un organismo costituzionalmente stabilito che non riusciamo a far uscire dal limbo della irrilevanza e della inconsistenza. Non vogliamo affrontare un dibattito serio sul futuro e sul ruolo di questo istituto rappresentativo del pluralismo sociale nel modesto scenario rappresentativo e decisionale del nostro ordinamento democratico costituzionale, ma intanto facciamo finta di garantirne la rivitalizzazione attribuendogli funzioni da bibliotecario, cioè da raccoglitore di documenti, di contratti collettivi, di promotore di indagini, e di relazioni, che rischiano di non essere né adeguatamente consultate, né acquisite al patrimonio decisionale di chi poi deve fare le leggi. Ritengo che dobbiamo uscire da questo rito e da questo malvezzo. rito e da questo malvezzo. In questa stagione sedicente orientata alle grandi riforme dobbiamo affrontare il ruolo e lo spazio del pluralismo sociale rappresentativo in una moderna democrazia in cui il pluralismo politico e partitico non esaurisce la ricchezza del pluralismo di una società contemporanea evoluta come la nostra. Dobbiamo pertanto superare il malvezzo di continuare a caricare

e senza la dovuta meditazione rilancia in modo disordinato la funzione del CNEL, ma occorrerebbe entrare seriamente nell'ordine di idee di una riforma costituzionale che elimini tale organo. È un organo costoso, della cui utilità si discute ormai da decenni, senza che si sia mai arrivati a definirne un compito congruente rispetto all'assetto attuale delle nostre istituzioni. Mi sembra che ancor meno esso avrà una funzione congruente con l'assetto federale che ci proponiamo di costruire per la Repubblica. ma non rivitalizzarlo. L'Italia ha bisogno di individuare tutti i rami secchi, tutte le strutture che non servono e che possono essere eliminate, soprattutto quando si tratta di strutture

«Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali

La prima è stata accennata ieri da esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Mi è difficile accettare che di un organo, che è comunque di carattere giurisdizionale, possano far parte rappresentanti nominati dalla politica, dal Consiglio regionale o dal Consiglio delle autonomie, che è poi la riunione di politici che provengono dagli enti locali.

La seconda obiezione, se permettete, è che, nella carenza ormai del sistema dei controlli, che sono stati largamente smantellati,

che vanno ad essere controllori dei propri solidali di partito o di corrente negli atti amministrativi deliberativi che essi pongono in essere, è un bel colpo alla credibilità di questo organismo di controllo; ne mette a rischio la credibilità e va a smantellare, a sbrecciare quello che dovrebbe essere un presidio, per quel ne che ne resta, di controllo sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Questo mi mette sinceramente in seria difficoltà. Questa norma è stata introdotta dai colleghi della Camera e con tutto il dovuto rispetto me ne rincresce. Non ne faccio una questione decisiva sul voto del provvedimento che dobbiamo sostenere, portare avanti e anzi licenziare senza navette, che a questo punto sarebbero non giustificate;

Già a dicembre del 2008 eravamo intervenuti per segnalare come sicuramente la Corte dei Conti necessiti di una riforma, che però deve essere organica, seria ed approfondita, e invece l'articolo conteneva e contiene al proprio interno delle norme contraddittorie tra di loro, che sono sicuramente insufficienti a soddisfare le esigenze non soltanto

non potrebbe essere realizzata con un emendamento e soprattutto all'interno di un collegato alla finanziaria. Qui ricordavamo, e ricordo ancora rapidamente, come venga modificata la coerenza del sistema costituzionale di controllo esterno della Corte dei conti, controllo che innanzitutto verrebbe ad essere asservito e subordinato ai governi centrali e locali e ciò, sottolineo, a detrimento in particolare del corretto rapporto che deve esistere con il Parlamento e quindi con queste Assemblee elettive. Peraltro, questo comma 4 dell'articolo 11 introduce una modifica ulteriore, che è quella di una previsione di nomine di natura politica all'interno di un ordine giurisdizionale. Qui è evidentissima - ed è stata sottolineata anche ieri nelle fasi preliminari e in sede di questione

Crediamo che una situazione di questo tipo non possa essere assolutamente accettata, innanzitutto da un punto di vista costituzionale, ma anche nell'ottica della trasparenza,

è in contrasto anche con il buon senso. Introduciamo all'interno di una magistratura simpatici signori che, oltre ad essere nominati dai controllati, veste di magistrati a tutti gli effetti e quindi entrano in un organo giurisdizionale senza alcuna forma di concorso, per cooptazione politica.

ma poi si impone - e non sappiamo se la norma è costituzionale anche sotto questo profilo - un onere a carico delle Regioni: lo Stato chiede alle Regioni di effettuare nomine impone alle Regioni medesime di pagarne i costi. Riteniamo che questa norma vada assolutamente abrogata, perché non ne riusciamo a comprendere neppure lo spirito politico, se non quello di creare*...

Stavo dicendo che anche sotto il profilo politico questa norma introduce grande confusione in un organo che è contemplato nella Costituzione e che è regolato

per sottolineare la contrarietà più convinta dell'Italia dei Valori alla distorsione a cui va incontro la Corte dei conti. Il Governo negli ultimi tempi ha La Corte dei conti dovrebbe essere un organo di autogoverno, che non può subire interferenze da parte dell'Esecutivo. Invece, si mettono in essere misure che garantiscono di fatto la possibilità per l'Esecutivo di interferire con questo organo giurisdizionale. Siamo in una dimensione di alterazione costituzionale.

che in realtà è stata abrogata soltanto un anno fa con la legge finanziaria dell'ultimo Governo Prodi, approvando un maxiemendamento che conteneva di tutto e di più, quindi anche l'abrogazione di questo sistema che è rimasto in vigore nel nostro Paese dal 2003 al 2008.

spezzoni e lacerti di tentativi di semplificazione che ridondano all'interno di altre leggi. Credo che alla fine ciò produrrà una complicazione e probabilmente prima o poi il Parlamento ne dovrà prendere atto.

uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della relativa contrattazione collettiva, prevedendo, tra l'altro, la tendenziale assimilazione della disciplina a quella relativa al lavoro privato, in particolare in materia di relazioni sindacali, promuovendo l'efficienza delle procedure di contrattazione collettiva, la previsione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, promuovendo meritocrazia meritocrazia e misure premiali, a fronte di un maggior rigore nella valutazione della responsabilità dei dipendenti, valorizzando altresì il principio di concorsualità ai fini dell'accesso al lavoro pubblico e delle progressioni in carriera. Sebbene il Gruppo UDC, SVP e Autonomie ne condivida le finalità, il provvedimento non può meritare un voto favorevole, sia perché concede un tempo troppo ampio al Governo per l'attuazione delle deleghe, in contraddizione con la natura di un disegno di legge collegato alla finanziaria, sia perché presenta alcuni elementi di criticità. Il percorso del provvedimento che stiamo per approvare era stato annunciato con grande enfasi e si era intravisto un obiettivo, che sembrava aderente alle aspettative

il fulcro per la lotta agli sprechi, per la riduzione della spesa pubblica, per l'innovazione, per il rapporto di efficienza, per la valorizzazione del merito, per la responsabilità dei dipendenti, per l'assenteismo e il controllo sulla scarsa produttività, che il Ministro ha chiamato «lotta ai fannulloni». Ci saremmo aspettati una partecipazione diversa da parte del Governo. Una partecipazione dinamica rispetto alle proposte avanzate, sia nelle Commissioni sia nell'Aula del Senato. Il Governo anche in questa occasione ha dimostrato poco rispetto per il Parlamento. Riforme di così rilevante portata o si fanno con il contributo di tutti o o sono riforme ridotte, che rimangono solo sul piano progettuale, senza esplicitarsi ed attualizzarsi. Signor Ministro, ci manca una valutazione complessiva e generale, con riferimento al problema della dirigenza generale, con tutti i problemi che abbiamo avuto abbiamo avuto e che ci trasciniamo, dalla separazione tra la responsabilità del potere politico e quella della dirigenza amministrativa, in un momento in cui lo Stato perde alcune sue attribuzioni per effetto del ruolo sempre più predominante delle Regioni e delle autonomie locali. Ci manca anche il coinvolgimento del Parlamento, nonché il dialogo e la possibilità per noi senatori di dare un contributo legislativo per formare un testo più completo. Per tali ragioni, annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

per non essere d'accordo con questo provvedimento. Li elenco, cercando di farlo con la massima semplicità: il primo punto riguarda l'assoluta contrarietà nei confronti delle disposizioni relative alla questione della Corte dei conti, su cui ci siamo intrattenuti appena poco tempo fa. Si assiste ad una distorsione di un organo che dovrebbe essere indipendente; lo si rende meno indipendente, suggestionabile da parte dell'Esecutivo ed in questa maniera si incrina quel tipico meccanismo di controllo reciproco che funziona quando funziona la democrazia. Questo tipo di soluzione adottata per la Corte dei conti, in realtà, non avrebbe dovuto essere introdotta in questo provvedimento. Più ne fosse stata fuori, più ne avrebbe guadagnato la chiarezza della legge. Il secondo punto riguarda la perplessità intensa relativa alla logica con cui l'attività legislativa finisce per prevalere sulla contrattazione collettiva. è una progressiva intenzione di ridurre gli spazi della contrattazione collettiva e di sottoporne

Questo cela in sé un rischio immanente ed è il fatto che, se si adotta questa logica, qualsiasi legge o leggina di carattere settoriale, magari spinta da interessi particolari, da pulsioni corporative, può infilarsi nella normativa di carattere generale e determinare una distorsione anche di natura finanziaria. Si potrebbe assistere ad un meccanismo per cui, derogando per norma la potestà contrattuale, all'interno di questa opera di deroga alla rovescia, si insinuino pulsioni corporative ed anche una certa tendenza - lo prevediamo con facilità - all'incremento di spesa. Il terzo punto di contrarietà riguarda il modo particolare con cui è stato creato l'organismo centrale con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio dei dipendenti ed alle funzioni di valutazione. Mi sono già trattenuto su questo argomento illustrando un emendamento. La preoccupazione è questa: tale organismo, che dovrebbe essere dipendente, rischia di non esserlo perché sarà di fatto di nomina governativa e per di più è straordinariamente costoso. Fatti i conti, siamo di fronte ad una spesa prevedibile di circa 10 milioni di euro per cinque componenti, i quali avranno magari anche la più straordinaria professionalità, però, francamente, mi sembra ci sia una sproporzione tra l'esiguità della commissione dell'indagine e la spesa. Penso che si possano temere, di fronte a questo contesto, le premesse per la costruzione di una cosa che è tutt'altro che omogenea all'aspirazione della semplificazione.

anche avere soltanto questa fantasia, prodotta però dalla lettera delle cose, nei confronti di un'entità che invece doveva essere fin dall'inizio l'emblema della chiarezza, della trasparenza e della visione sgombera di interessi particolari. Il quarto punto di contrarietà riguarda l'argomento su cui si è intrattenuto il collega Lannutti a lungo: mi riferisco agli inceppi che vengono messi tra i piedi della cosidetta *class action,* che io preferirei chiamare azione collettiva. Nei confronti di essa vi sono essenzialmente due elementi che fanno riflettere:

per cui - una volta che questa difficile, complicata, inceppata azione collettiva sia arrivata a compimento si può arrivare perfino alla punizione del pubblico dipendente colpevole ma si esclude in modo sistematico il risarcimento del danno. la cosa appare contraddittoria con le intenzioni stesse dell'azione collettiva. I cittadini sprecano iniziative, soldi, impegno personale, per costruire una cosa difficile come la rappresentazione degli interessi dei cittadini in un organo collettivo informale, di fronte all'autorità dell'amministrazione; si danno da fare, attraversando un *iter* complicato

dell'ultimo emendamento - è costituito dal fatto che anche in questo provvedimento, che ha una sua serietà, viene introdotta per così dire di sbiego una parte dell'iniziativa di semplificazione. Per tutti questi motivi, l'Italia dei Valori vota contro.

si è sempre battuta con l'obiettivo di avere comunque una pubblica amministrazione efficiente: diritti ai pubblici lavoratori ma con efficienza. tutti ormai sul fatto che sia fondamentale attuare politiche di rinnovamento di una pubblica amministrazione quasi sempre percepita come lenta, costosa e inefficace. È quello che prospetta questo importante disegno di legge delega, a cui si è giunti attraverso un contributo costruttivo da tutte le parti di entrambi i rami del Parlamento, Senato e Camera. quindi di un testo per lo più condiviso, volto alla razionalizzazione dell'amministrazione pubblica cercando di massimizzarne la produttività, in un'ottica di meritocrazia e valorizzazione del dipendente, cercando nel contempo di migliorare l'offerta di beni e servizi pubblici messi a disposizione del Paese. Per fare ciò si prevede il mercato del lavoro pubblico converga verso quello del lavoro privato. Si sono stabiliti, inoltre, criteri direttivi relativi ad un nuovo approccio della disciplina sulla valutazione delle strutture e del personale della pubblica amministrazione. Si prevedono, infatti, nel testo del provvedimento in esame misure finalizzate a premiare i dipendenti meritevoli e a far scattare sanzioni nei confronti di quei dirigenti che non c'entrano gli obiettivi prefissati per l'attività dei loro uffici,

A tale proposito, vorrei soffermarmi sull'importanza dell'introduzione del principio teso a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni di accedere direttamente alle informazioni relative alla valutazione del personale, oltre che della previsione

introdotti meccanismi premiali per quelli meritevoli - lo abbiamo già detto -, prevedendo che parte delle economie derivanti dai risparmi sui costi di funzionamento e destinati al personale coinvolto dal processo di ristrutturazione e razionalizzazione siano attribuiti in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e per contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo. Riguardo al contrasto del fenomeno dell'assenteismo, da parte di questo Governo, si sono già attuati diversi interventi decisivi ed incisivi che hanno dato i suoi frutti, soprattutto per ciò

che oggi si fa sul serio e che non si deve sgarrare. Questi dati, infatti, hanno evidenziato come queste misure devono aver indotto comportamenti più corretti e responsabili

riguardante la previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando come titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico. Tali criteri sono destinati a favorire l'ottimizzazione del lavoro pubblico e, in particolare, ad evitare che, come spesso accade, i vincitori di concorso in Regioni diverse da quelle di residenza chiedano immediatamente il trasferimento, compromettendo così le esigenze funzionali del sistema pubblico. Quello che la nostra gente vuole è poter contare su una pubblica amministrazione moderna ed efficiente che possa chiaramente rappresentare

le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e gli stipendi sono sempre e comunque limitati allo stretto indispensabile.

ho sempre sostenuto che pubblico non sempre è peggio di privato; quindi, la filosofia del provvedimento è quella di aver sempre un pubblico efficiente, migliore, trasparente, veloce e, pertanto, noi come Gruppo della Lega Nord siamo convinti che dalla presente riforma

per migliorare i provvedimenti. Rivendichiamo pienamente tutte le parti, anche innovative, che insieme abbiamo costruito e che fanno parte della nostra proposta di legge, che in particolare sottolineavano i punti riguardanti l'innovazione della pubblica amministrazione, l'efficienza, il merito, la trasparenza, la valutazione. Su questo terreno, signor Ministro, la sfida è molto alta e noi la sfidiamo ancora di più. Il Partito Democratico è convinto che la pubblica amministrazione sia un vero fattore di sviluppo e di competitività del Paese. È infatti per noi un elemento di arretratezza rispetto ai Paesi d'Europa

rispetto ai compiti di *governance*, sempre più complicati, rispetto alla presenza di tanti attori sociali, s'impone ai decisori politici la necessità di un'amministrazione qualificata, competente e che sappia reggere a queste sfide.

di lavorare per obiettivi, di tendere a dare risposte ai cittadini e all'impresa. Efficienza, quindi, produttività, merito, trasparenza: queste le proposte del Partito Democratico, che non si è sottratto ad un confronto di merito, che ha lavorato sull'obiettivo, come enunciato anche nella proposta del Governo, di una convergenza sui temi del lavoro pubblico e del lavoro privato; ma anche sottolineando attentamente che la pubblica amministrazione non è un'impresa. Essa ha bisogno di alcuni cardini, di alcuni fondamenti, perché sia veramente esercizio anche della funzione democratica nella sua ossatura e nella sua dirigenza, al di là delle maggioranze che si possono avvicendare. Per questo, signor Ministro, non ci ha convinto il primo approccio, l'impianto iniziale con cui era stato presentato questo provvedimento - al di là delle declamazioni, delle sue affermazioni

Possiamo pensare che si potrebbe produrre una confusione. Ci auguriamo, e lavoreremo a tal fine, che nelle norme attuative questi aspetti siano chiariti e non si torni assolutamente indietro. Sia chiaro, non è che non vediamo le degenerazioni di alcuni aspetti della contrattazione decentrata, come le rendite di posizione o i corporativismi. Il Partito Democratico raccoglie la sfida, va più avanti, ma sicuramente lei ci voleva proporre, e rischia di proporre anche con questi emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, un rimedio peggiore del male. Una legge che ritorna a prevalere sulla contrattazione, una politica invadente che si introduce in un rapporto che non le è proprio (dovrebbe soltanto tracciare le linee, le cornici); la possibilità ancora una volta di tornare a maggioranze che possono di volta in volta alternarsi e che usino la pubblica amministrazione come camera di compensazione, magari anche in tempi di elezioni. Se c'è stato un guaio nel nostro Paese è proprio questo, che la classe dirigente non ha affidato una funzione e una missione alla pubblica amministrazione, che non ha creato una schiera di dirigenti pubblici all'altezza dei tempi e delle sfide, che ha usato invece la pubblica amministrazione perché fosse non competente, non qualificata e quindi più prona ai *desiderata* dei decisori politici. Insomma, lo spirito del decreto legislativo n. 29 del 1993 tenta ancora invano e con difficoltà di affermarsi. Questo quindi è un nostro terreno di sfida, signor Ministro, per cui riteniamo addirittura, per quanto apprezziamo i passi avanti, insoddisfacente il percorso fatto fin qui. lei, in quanto rappresentante del Governo - non si tratta di una notazione personale - ha scelto di parlare della pubblica amministrazione in modo un po' riduttivo, ritornando quasi sui singoli comportamenti dei lavoratori come se questi, e non i temi che ho tentato di argomentare, fossero il male della pubblica amministrazione. Ecco, noi ribadiamo il rigore, il merito ma non la compressione dei diritti. Siamo per uno sguardo responsabile e qualificato sulla pubblica amministrazione; siamo per unire le forze del lavoro, siamo per la pazienza di chi governa, che per produrre riforme deve sfidare anche la composizione del consenso. Siamo per un processo innovativo della pubblica amministrazione; non si tratta solo di investire risorse finanziarie. Ecco, lancio qui una sfida: perché non iniziare un processo di riforma vero di tutta la pubblica amministrazione, connettendosi alle università, a tanti centri di eccellenza pubblici e privati che su questi temi hanno lavorato, e fare della funzione pubblica un vero motore di una sperimentazione che si avvia in tante parti del Paese, supportandola ed aiutandola, così come abbiamo detto noi nella nostra proposta sui temi della valutazione? Signor Ministro, la campagna mediatica che lei ha voluto stabilire lascia una traccia che ci mette anche molto in difficoltà, nonostante gli apprezzamenti e nonostante il lavoro fatto in comune. Chiediamo un quadro più generale di valutazione, al di là dei punti controversi che rimangono su questo provvedimento

smetteranno di svolgere le proprie funzioni. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori; non vogliamo utilizzarli come ammortizzatori sociali ma decidiamo quale vuole essere la linea di azione. Siamo pronti sempre ad una collaborazione attenta, puntuale e di qualità su questi temi; non ci sottraiamo e non ci siamo sottratti, ma per le motivazioni più generali di peggioramento del provvedimento e per quelle che ho tentato di argomentare voteremo contro, a lavorare e a collaborare in tutte le fasi di attuazione dei procedimenti che seguiranno e degli altri provvedimenti che lei porterà nelle Commissioni.

signor Ministro, onorevoli colleghi, la riforma della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico, che quest'Assemblea si appresta ad approvare, è una riforma vigorosa e intensa. è una riforma vigorosa e intensa. I dati ormai acquisiti nella letteratura scientifica internazionale individuano una relazione di questo tipo: ogni dieci punti di produttività del lavoro pubblico

che questa riforma è in grado di recuperare a regime non meno di 20 punti di efficienza del fattore lavoro della pubblica amministrazione, e più probabilmente si orienta ed indirizza a conseguirne 30, allora è evidente che siamo in presenza di una riforma dal significato economico imponente per l'intero sistema economico del nostro Paese. Questa positiva imponenza, questa straordinaria capacità di mobilitazione dello sviluppo acquisisce un ruolo ancor più cruciale ora che la grande crisi ha fatto alluvionale irruzione mettendo davvero in difficoltà l'intera articolazione del nostro sistema economico. È decisivo che vengano sottratte risorse per essere virtuosamente destinate al sostegno nel nostro sistema industriale dei servizi aperti, prelevandole da quella pubblica amministrazione che viene sempre percepita - e non irragionevolmente come zavorra, come ostacolo, come impedimento al pieno dispiegamento della capacità di generazione competitiva del nostro sistema. Questo trasferimento di risorse da una pubblica amministrazione pesante, opaca, occlusa, al sistema delle imprese, impegnato in una lacerante competizione nell'arena internazionale, può diventare un elemento decisivo per superare il deserto della crisi e per riapprodare felicemente in una condizione di positività economica. La chiave della riforma che stiamo per approvare è l'introduzione massiccia e scandita del principio di responsabilità nella pubblica amministrazione, trasformando quel principio, trasformando quella cultura in una prassi. Non è un caso che mi permetto di sottolineare come tra l'altro quello stesso principio, quella stessa cultura e quella stessa prassi della responsabilità siano il complessivo vettore ideologico - se mi perdonate l'espressione - della riforma sul federalismo fiscale

l'introduzione della cultura della responsabilità è quello dello spostamento netto del baricentro della configurazione organizzativa della macchina pubblica dal procedimento al provvedimento, cioè il sistema passa un'organizzazione autoreferenziale concentrata e incentrata sulla propria mera sopravvivenza, per recuperare invece la pienezza della relazione con lo scopo per il quale una pubblica amministrazione è stata costituita e istituita. C'è questo recupero dell'orizzonte di senso che legittima la pubblica amministrazione ad essere tale, ponendola in una relazione fertile con i cittadini i clienti. Proprio questo nuovo nesso di sostanzialità per cui il centro è il provvedimento, per cui il centro è lo scopo per il quale la macchina amministrativa esiste, davvero dà un segno forte verso il recupero di quei segmenti, di quegli spezzoni spesso così densamente raggrumati di antipolitica, che sono uno fra i grandi pericoli che il nostro Paese corre, laddove non riesca a restituirli a compiutezza, di rientro in un'autentica logica democratica. Una buona riforma della pubblica amministrazione è decisiva per dire agli italiani che la politica è buona e dunque essa non va respinta, ma va praticata, va attraversata con consapevolezza e con partecipazione. *(Brusìo).* PRESIDENTE. Colleghi, Colleghi, per favore, consentite al senatore Castro di terminare la sua dichiarazione di voto. CASTRO *(PdL)*. La ringrazio, signora Presidente. Bill Clinton ed Al Gore nel lanciare il loro grande programma «reinventiamo l'amministrazione» (mi astengo dall'espressione inglese perché ho assunto l'impegno con il presidente Nania di non ricorrere ad alcuna espressione espressione della *koinè* manageriale internazionale e credo che anche con la presidente Bonino valga lo stesso impegno). Quindi «reinventiamo l'amministrazione» in qualche modo è anche il segno che connota la riforma che oggi ci apprestiamo ad approvare. I tratti fondamentali possono ulteriormente essere riassunti in un recupero marcato di efficienza lungo una linea che va ribadita con chiarezza anche alla luce di talune piccole polemiche che si sono recentemente fatte segnare. Finalmente si sconfigge il principio, nel nostro Paese troppo volte malamente recitato, che poche risorse e buona qualità non riescano ad andare d'accordo. L'efficienza, intesa come cultura nemica dello spreco, è portatrice di per sé di buona qualità. Usciamo, per cortesia, da questa mitologia tanto più ingenua quanto più in realtà ipocrita, secondo la quale solo dotazioni generose di risorse possono determinare buona qualità per i clienti cittadini. È vero esattamente il contrario: tutte le buone esperienze italiane ed internazionali, anche nel settore privato, persino nel segmento del lusso, dicono che più feroce è la caccia allo spreco, più alta è la capacità di generazione della qualità nel processo e nel prodotto. Un sì netto anche alla meritocrazia, con l'intelligente equilibrio secondo il quale il merito che viene ricercato, riconosciuto e remunerato non è soltanto il merito individuale, del singolo funzionario, ma è il merito di un'organizzazione, di una squadra, che viene organizzata dal dirigente al quale viene affidata una strumentazione efficace per condurre quella squadra alla pienezza dei suoi risultati. Profonda è anche la riforma nella direzione del cambiamento della cultura delle relazioni industriali nella pubblica amministrazione, che programmaticamente ed intensamente passano dal vecchio, stantio modello consociativo ad un modello partecipativo che rende queste stesse relazioni industriali nel pubblico impiego compiutamente coerenti con le riforme in atto nel settore privato.

una piena convergenza, una compiuta confluenza del voto del Partito Democratico su questa riforma. Ho l'impressione, e lo dico con personale rammarico, che un voto contrario

più attento alle diverse articolazioni organizzative, agli orizzonti più efficaci delle esperienze internazionali di quanto non fosse all'ingresso in Parlamento. Lo stesso lavoro intelligente, competente, attento del presidente Vizzini, che è stato un magnifico relatore, corre forse il rischio di essere vanificato. Non voglio però ascoltare le voci di quei commentatori, di quegli spagirici, tanto più perfidi quanto più pessimisti, che vogliono vedere in questa decisione del Partito Democratico una sorta di regressione barbaricamente clanica intorno ad un grumo identitario e conservatore; no, non sono assolutamente d'accordo su questa interpretazione: credo sia semplicemente

ritiene davvero significativa l'apertura fatta dal ministro Brunetta nel momento in cui ha dichiarato di mantenere intatto un percorso ad alta densità partecipativa nella emanazione dei decreti delegati, quel ministro Brunetta che esce in qualche misura dalla decisione del Partito Democratico rafforzato come un nitido riformatore, capace di intelligenza e di energia. C'è un filo rosso che collega il giovane Brunetta

quella che oggi esce dal Senato è una riforma che consentirà fra qualche anno alla pubblica amministrazione italiana di essere, come il settore dell'auto sportiva, come quello dell'aeronautica, come quello dell'elettrodomestico, come il sistema della moda, come il sistema della gioielleria, una grande eccellenza italiana.

Calma, colleghi. Facciamo le opportune verifiche e non chiudiamo la votazione fin quando non sono stati effettuati gli opportuni controlli.

Signor Presidente, il provvedimento che andiamo ad esaminare

questo contiene varie misure che si riferiscono allo sviluppo economico, alla semplificazione legislativa ed amministrativa, alla competitività, nonché altre misure in materia di processo civile.

non sono però per questo meno importanti, proprio ai fini che si propone questo disegno di legge, vale a dire quelli dello sviluppo economico, della competitività e della semplificazione.

quanto riguarda il contenuto delle singole parti di questo provvedimento - mi occuperò qui della parte di maggiore competenza della Commissione affari costituzionali l'articolo 1 contiene provvedimenti per gli interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate atti a facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Si tratta di una norma molto importante perché, proprio in quelle aree del Paese, è importante che ci sia uno

altresì che ogni rinvio ad altre norme indichi in forma integrale o sintetica il testo o la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento. Si tratta di princìpi generali che vanno applicati sempre dal Governo quando redige testi legislativi.

delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, lasciando che le altre invece vengano cancellate secondo le norme che abbiamo già discusso in altra sede.

categorie di leggi che è necessario restino in vigore. Contiene poi norme per coordinare questo intervento con le altre normative in vigore sul merito. merito. L'articolo 3-*ter* attiene a modifiche alla disciplina dei regolamenti e dei testi unici compilativi. Si tratta di una misura analoga a quella degli articoli precedenti, ma riferita a questa particolare fattispecie. L'articolo 4 reca misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, così da adattarli alle nuove esigenze e da superare diseconomie che impedivano nel passato, ad esempio, a certe strutture, di espandere la propria attività nel rilascio di autorizzazioni, visti e documenti di competenza, anche quando queste avrebbero recato maggiori introiti, introiti, anziché maggiori oneri. Si tratta di dare maggiore autonomia e maggiore semplicità nelle procedure.

efficacia. L'articolo 7 interviene sulla Conferenza di servizi e sul meccanismo del silenzio assenso. È importante che in questo articolo sia stata introdotta la previsione circa la partecipazione, senza diritto di voto,

si occupa della tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali. L'articolo 9, di molto ridotto nel suo passaggio in Commissione a causa della eliminazione

per realizzare ed individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria presso le farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È una norma molto importante e vicina ai cittadini, a differenza di altre che restano spesso nell'ambito della pubblica amministrazione, pur esplicando i suoi effetti ben al di fuori di essa, perché si prevede che le farmacie possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto dell'attività del

L'articolo 9, come dicevo, si propone di far partecipare le farmacie al servizio di assistenza domiciliare a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche per garantire il corretto utilizzo dei medicinali; di collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione; di realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale; di consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici. Tutte queste attività andranno remunerate entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il Servizio sanitario nazionale. Questo è un principio che viene usato in diverse parti della normativa introdotta da questa legge. di cui si occupa l'articolo 9 è una semplificazione a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, simile a quella che si offre ai cittadini; questi Comuni, nel caso in cui vengano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti e provvedimenti o copie dei medesimi o documenti consimili, possono semplicemente limitarsi a citare qual è la pubblica amministrazione presso la quale quei documenti sono reperibili, in modo da non caricare gli oneri di ricerca di archivio sui Comuni stessi, che hanno un personale ridotto date le loro ridotte dimensioni. Sono stati invece stralciati altri provvedimenti che riguardano i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che potranno essere, con opportune rivalutazioni, esaminati in altra sede, ad esempio nel codice delle autonomie. l'articolo 9-*bis* che prevede un differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale. L'articolo 10 prevede modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale, prevedendo la priorità per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina

con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato disoccupazione a causa della crisi economica. introduce misure per la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate. L'articolo 11-*bis* interviene sul Fondo nazionale di garanzia. L'articolo 12 introduce misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale.

interviene sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale del turismo. L'articolo 13 è stato soppresso dalle Commissioni. L'articolo 14 introduce misure per la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti, inclusi i segretari comunali e provinciali, e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

L'articolo 16 è stato stralciato, così come il successivo articolo 17. L'articolo 18 si occupa della diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e dei tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico. L'articolo 20 contiene disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari. L'articolo 21 si occupa della tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. si occupa dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea incoraggiando l'uso dello strumento informatico, pur con misure che salvaguardino coloro che da questa pubblicazione traevano un giusto beneficio. 23 introduce alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale, allo scopo di rendere questa tecnologia sempre più efficace ed impiegata positivamente nella pubblica amministrazione; lo stesso tema è trattato dall'articolo 23-*bis*. L'articolo 24 si occupa ancora di tecnologia avanzata, in particolare del sistema cosiddetto VOIP (Voce tramite protocollo Internet) e del sistema pubblico L'articolo 24-*bis* modifica la Carta nazionale dei servizi. L'articolo 25 prevede la riallocazione di alcuni fondi. L'articolo 26 introduce misure a favore del risparmio energetico. Dopo l'articolo 26 sono stati introdotti alcuni articoli importanti: il 26-*bis* contiene disposizioni all'Avvocatura dello Stato e in esso vengono modificati i criteri di ripartizione dei proventi di determinati tipi di cause;

del federalismo, contiene una clausola di salvaguardia riguardante le Regioni a Statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano. Questi ultimi articoli non sono stati modificati in Commissione.

sì che il giudizio civile abbia una durata consona alle attese dei cittadini che al giudice civile si rivolgono. Ho l'idea che la parte normativa abbia una sua importanza, però ritengo anche che coloro anche che coloro che si occupano concretamente del processo civile non possano essere ritenuti del tutto al di fuori dei problemi di

c'è un numero eccessivo di avvocati; questo comporta che il numero delle cause sia notevole e che le possibilità di conciliazione diminuiscano.

sono stati accolti emendamenti provenienti da tutte le parti. Sono oltre 20 gli emendamenti del Governo, della maggioranza e dell'opposizione che riguardano le norme di cui ci stiamo occupando.

le decisioni su questa materia non devono più essere delle sentenze, ma solo delle ordinanze. Successivamente, per quanto riguarda le sentenze, molto opportunamente si dice che nella sentenza non è più necessario

Anche nello svolgimento degli incarichi, i consulenti, i custodi e gli altri ausiliari devono rispettare i termini fissati dal giudice che, secondo questa norma, non devono superare i tre mesi, salvo casi che devono essere ritenuti eccezionali e, quindi, motivati dal giudice che assegna il termine. Se il consulente, il custode e gli ausiliari del giudice non rispettano questo termine la sanzione è la revoca

Per quanto riguarda le memorie, di cui all'articolo 183, mentre prima la norma diceva che il giudice deve concedere il termine per le memorie difensive, adesso può concedere

la procedura relativa alle consulenze. Uno dei punti importanti di questa decisione è la testimonianza scritta. è la testimonianza scritta. Nel testo della Camera si diceva che il giudice, sentite le parti, poteva chiedere che i testimoni rispondessero ai quesiti non presentandosi davanti al giudice stesso ma compilando un modulo, che dovevano fare autenticare da un segretario generale e poi consegnare.

che non si tratti di documenti di spesa (fatture di incidenti stradali o di altro genere); in questi casi il teste rilascia all'avvocato che lo ha dedotto come teste la deposizione scritta e l'avvocato la presenta

Un altro punto centrale della riforma è il cosiddetto filtro, vale a dire l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. questa nuova disposizione: «Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza

Nella norma vengono indicati in dettaglio e con precisione tutti i casi di ammissibilità, non è cioè una norma di carattere negativo che dice quali ricorsi non sono ammissibili, ma vengono indicati con esattezza i casi di ammissibilità. Tra questi, nella prima versione approvata dalla Camera, c'era la cosiddetta doppia conforme: se la sentenza di primo e secondo grado fossero state identiche, non era ammissibile il ricorso per Cassazione. del Governo, è stata esclusa perché tutti abbiamo convenuto sul fatto che due errori non fanno una verità, due sbagli non danno luogo ad un'interpretazione corretta. Viene snellito anche il procedimento del pignoramento presso terzi e si inserisce il procedimento sommario di cognizione, quale prevede che la domanda sia proposta non già con citazione ma con ricorso. Però, tutto va bene solo se il giudice che riceve il ricorso fissa la prima udienza in termini brevi;

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno

una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili. Come molti dei senatori sanno, sono stati inseriti diversi procedimenti civili

che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale». noi relatori, il senatore Malan ed io, abbiamo presentato all'Assemblea un emendamento per far sì che il cosiddetto rito societario, che è entrato in vigore qualche anno fa e che non funziona assolutamente, venga abolito, salvo ovviamente che per i procedimenti in corso. Sempre al fine di ridurre la durata dei procedimenti, viene data al Governo un'ulteriore delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. prima che inizino i giudizi deve essere fatta questa mediazione con tutta una serie di regole, che sono esposte e ben dettate nell'articolo 39 che è stato approvato.

tra lo Stato e l'amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo, come tutto il resto, sulla durata dei processi.

*(PD)*. Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, come Partito Democratico abbiamo presentato tale questione sospensiva in relazione al disegno di legge in esame perché esso solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito, che non sono superate dall'esame che abbiamo effettuato all'interno delle Commissioni 1a e 2a. All'interno di queste Commissioni, si sono anzi verificate continue presentazioni di emendamenti, accavallamenti a non finire, contraddizioni, accelerazioni e frenate, e abbiamo assistito a contrasti, anche pesanti, tra la maggioranza e lo stesso Governo. Per quanto riguarda in particolare i profili metodologici, non si può in alcun modo condividere la scelta di introdurre una così incisiva riforma del codice di rito civile del 1942 nell'ambito di un collegato alla finanziaria, esaminato in tempi ristretti, non certo adeguati alla portata delle innovazioni ordinamentali previste, in assenza della organicità, sistematicità e completezza che sarebbero necessarie per ogni riforma. Basti pensare, in proposito, come il disegno di legge in questione non preveda disposizione alcuna in merito ad una delle fasi del processo civile, quale la fase esecutiva, che rappresenta invece una delle parti maggiormente meritevoli (se non addirittura bisognose) di riforma, così come rilevato dalla sensibilità degli operatori del settore e dagli utenti della giustizia. modo, un'altra questione, quella relativa all'accelerazione dei vari momenti processuali, non è stata adeguatamente approfondita ed affrontata. Questo rilievo è *a fortiori* asseverato dal fatto che una delle parti maggiormente innovative della riforma proposta, ovvero l'unificazione dei riti del processo civile, è stata introdotta soltanto con un emendamento, sulla cui opportunità non è stato possibile acquisire specifici e aggiornati pareri di avvocati, della magistratura, di docenti ed esperti in materia, degli operatori del settore, pareri che ben avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo, a enucleare le reali problematiche del processo civile, e soprattutto della sua fase esecutiva, che solo chi pratica ogni giorno le aule dei tribunali civili conosce davvero, nella loro complessità. Inoltre, l'emendamento in questione sull'unificazione dei riti, lungi dal dettare disposizioni autoapplicative (che avrebbero potuto essere previste in questo specifico settore), contiene invece una mera delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi in materia, peraltro secondo princìpi e criteri direttivi privi dei necessari requisiti di tassatività e determinatezza richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, soprattutto nella lettura fornitane da una consolidata

per l'emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; materia la cui delicatezza e complessità richiederebbe un approfondito confronto nel merito, merito, così come la materia fallimentare imporrebbe un confronto adeguato; confronto che invece non è reso possibile rispetto a meri principi e criteri direttivi, inseriti nel disegno di legge, che sono peraltro privi dei necessari requisiti anch'essi di tassatività e determinatezza richiesti dalla Carta costituzionale. Rappresento infine come esistano almeno tre disegni di legge di riforma completa del codice di rito processuale civile, disegni di legge d'origine sia della maggioranza che dell'opposizione, che si basano tutti sui lavori del comitato ristretto costituito nella precedente legislatura all'interno all'interno della Commissione giustizia (comitato ristretto presieduto dal senatore Caruso). I lavori avevano visto un'ampia condivisione, per cui le fasi conclusive di questi disegni di legge si possono ritenere non molto distanti tra di loro. Quindi, sarebbe davvero opportuno Per certi aspetti alcune parti di questa preannunciata riforma del processo civile rischierebbero di fare rivoltare nella tomba i nostri professori processual-civilisti.

Presidente, francamente siamo stupiti dalla presentazione siamo stupiti perché dall'inizio della legislatura da parte di tutte le opposizioni è stato imputato al Governo, quindi conseguentemente alla sua maggioranza, di interessarsi di problemi in qualche modo legati alla giustizia che però esulavano dal problema vero e fondamentale della giustizia italiana, cioè una giustizia dai tempi esageratamente lunghi.

si interessa di problemi non strettamente legati all'estrema lentezza della giustizia sia civile che penale, lentezza che rende invece necessario un intervento immediato. Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che nei due anni della precedente legislatura di parole ne sono state fatte tante, di commissioni anche, di risultati zero: questo è un fatto assolutamente incontestabile, perché è stata istituita una commissione ministeriale per la riforma del processo penale con risultato zero; è stata istituita una commissione per la riforma del codice penale con risultato parimenti zero. Si è detto che quello della giustizia è un problema gravissimo perché, anche se la lentezza della giustizia non occupa - così come non occupa - le prime pagine dei giornali e i resoconti televisivi, è altrettanto vero che la giustizia interessa milioni di italiani, tant'è che i processi pendenti sono 5,5 milioni. Si diceva che la lentezza della giustizia civile interferiva anche sulla competitività del sistema Italia, perché si diceva giustamente che molti investitori stranieri erano disincentivati a portare capitali in Italia stanti i ritardi clamorosi della giustizia civile. Ebbene, tra i primi provvedimenti messi in cantiere dal Governo, vi è stato anche quello della riforma della giustizia civile. Pensavamo che le opposizioni riservassero ben altro trattamento ad un'iniziativa che andava incontro non solo alle aspettative di tutte le opposizioni,

una riforma che incideva anche per una semplificazione - lo diremo più avanti - del sistema della giustizia civile. Una riforma tecnico-giuridica, non una riforma di sistema per la quale si prospettava una modifica costituzionale (non si parlava di una riforma che andava in qualche modo ad interferire sul Consiglio superiore della magistratura); una riforma che non toccava minimamente questioni delicate su cui immediatamente erano state erette barricate dalle opposizioni, e non solo da queste; posso riferirmi anche alla questione relativa alla separazione delle carriere

e subito dopo o subito prima la riforma della giustizia penale. Nel momento in cui il Governo ha posto mano in modo responsabile e con assoluta urgenza alla riforma della giustizia civile, noi ci siamo sentiti obiettare che si sarebbe dovuta seguire una strada diversa,

con particolare attenzione, come diceva prima di me il relatore, senatore Delogu, anche ascoltando (perché è importante ascoltare le opposte tesi dell'opposizione) e valutando positivamente tanti emendamenti di sostanza che sono stati prospettati dalle opposizioni e che sono stati recepiti dalla stessa Commissione e quindi dal Governo, c'è stata una particolare attenzione alle sollecitazioni che provenivano da parte dei colleghi dell'opposizione oggi possiamo dire tranquillamente che quella riforma che era stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento, oggi, così com'è uscita dalle Commissioni riunite, sia sicuramente una riforma migliore,

di alcune prospettazioni che ci venivano dal mondo della avvocatura: abbiamo ascoltato con attenzione gli avvocati ed anche i magistrati, che erano interessati alla riforma della giustizia civile e oggi si può tranquillamente dire che ci troviamo di fronte ad un testo non dico di gran lunga, ma certamente migliore rispetto a quello che era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Possiamo dire che una volta tanto il sistema bicamerale perfetto ha funzionato, questa volta, in questo ramo del Parlamento, stiamo per votare - e noi speriamo approvare - una riforma che certamente è da lungo tempo attesa contiamo possa trovare anche il consenso almeno di una parte delle opposizioni. Infatti, quando si parla di riforma tecnico-giuridica non dovremmo schierarci su posizioni ideologiche di maggioranza e di opposizione, di centrodestra e di centrosinistra, perché si parla di questioni tecniche rispetto alle quali non dovrebbero esservi particolari differenze.

Nel momento in cui si introduceva il giudizio sommario di cognizione, da parte di qualcuno, anche fuori dal Parlamento, giustamente era stato fatto osservare che si introduceva un nuovo rito. un nuovo rito. Nel campo della giustizia civile c'erano già troppi riti, per quale motivo se ne doveva introdurre uno nuovo? Era una considerazione che aveva una sua logica e una sua ragionevolezza, tant'è che abbiamo sollecitato il Governo il quale, proprio in base alle indicazioni dell'intera Commissione, ha presentato un emendamento volto a semplificare e ridurre drasticamente i tanti riti della giustizia civile.

era solo il giudizio di cognizione ordinaria. Poi, tempo dopo, venne introdotto il rito speciale del lavoro. C'era un solo rito, mentre oggi, colleghi senatori dell'opposizione, il vero dibattito è sul numero dei riti attualmente esistenti: c'è chi dice che sono 23, chi sostiene che siano 25 e chi 28. Con questo provvedimento finalmente si giunge ad una drastica riduzione dei riti, semplificando la vita non soltanto degli avvocati, ma anche dei magistrati, consentendo altresì una maggiore rapidità delle decisioni e mettendo la nostra giustizia finalmente sullo stesso piano, o quasi,